analogamente a quanto sta già accadendo alla Camera dei deputati su richiesta del mio collega, fatta pervenire al Presidente della Camera, per le vie brevi, nella serata di ieri.

mi permetto di formulare questa richiesta, affinché se ne possa discutere e possa essere accolta, nel solco della consuetudine parlamentare

Presidente, è prassi del Senato della Repubblica che se un Capogruppo chiede la convocazione della Conferenza dei Capigruppo questa gli venga concessa: quindi che ciò debba accadere anche in questa circostanza. Naturalmente non posso non sottolineare la necessità che le le scadenze, i termini e la continuità della nostra discussione sul disegno di legge costituzionale che precederà l'esame delle riforme non subiscano alcun rallentamento. Stiamo discutendo di una materia di grandissima rilevanza e di grandissima delicatezza.

Signor Presidente, anch'io credo che vada sottolineato il momento particolare che viviamo. Abbiamo iniziato nei giorni scorsi una lunga discussione che ha anche lo scopo di ricostituire un patto fiduciario tra le istituzioni e il Paese. Il senso del lavoro di questi giorni in fondo è questo, però il nostro è anche un Paese che ha bisogno di vedere le proprie tensioni ricondotte dentro un confronto civile e non ha bisogno di ulteriori momenti di esasperazione del confronto e del dibattito. concordo sull'esigenza di convocare la Conferenza dei Capigruppo; credo che tale richiesta debba essere accolta dalla Presidenza. Così come ha sottolineato il senatore Zanda, sin da questa settimana, ma anche dalla prossima, facciamo in modo che il calendario non subisca interruzioni nel prosieguo di argomenti importanti: oggi il disegno di legge costituzionale, la mozione sul nostro sistema di difesa e altri provvedimenti che sono in calendario. Credo che tutto ciò non debba subire dei ritardi. Quindi,

Sappiamo tutti quello che è successo in questi giorni. Il presidente Schifani ha chiesto tempo e la Lega Nord è d'accordo. Il PdL è uno dei maggiori partiti che sostengono questo Governo, quindi siamo perfettamente d'accordo che questi fatti debbano essere chiariti, e siamo d'accordo anche sulla convocazione urgente della Conferenza dei Capigruppo. [DE

il Parlamento, in questo caso il Senato, non credo debba nel modo più assoluto

Capisco la situazione complicata anche dal punto di vista politico, ma non credo che noi possiamo neanche lontanamente pensare di poter discutere anche solo la fissazione della data

non saremmo neanche i soli a non volere neanche lontanamente prendere in considerazione una tale ipotesi. Ieri abbiamo discusso molto, mi pare, dell'autonomia

dal senatore Schifani, ma ci permettiamo di ribadire come non sia impellente soltanto il lavoro prospettato dal senatore Zanda (e contro cui noi ieri abbiamo esplicitato le nostre posizioni, perché sulle riforme costituzionali sul tentativo di forzare la Costituzione il nostro no è stato abbastanza netto e chiaro): noi riteniamo che ci sia tanto altro da fare. Noi ci stiamo battendo affinché si restituisca centralità e pertanto dignità all'istituzione parlamentare. Era il senatore Tarquinio, quindi un senatore del Gruppo Pdl, che ieri rimarcava l'assoluta indifferenza con cui si svolgeva il dibattito; quindi colgo positivamente le parole della collega De Petris che ci invitava tutti nei fatti - e non soltanto nelle parole - a predicare ma poi anche a praticare la distinzione dei poteri, che è un fondamento del nostro ordine democratico. Ieri abbiamo saputo che un'importante agenzia di *rating* ha declassato il Paese, quindi penso che ci siano tante emergenze, e non soltanto

accolto sostanzialmente quella che è la celebrazione di una prassi, cioè di non opporsi alla richiesta di un Capogruppo di convocare una Conferenza dei Capigruppo. Con questo mio intervento, signor Presidente, intendo chiarire all'intera Aula che il mio Gruppo mio Gruppo ha votato convintamente la mozione che ha tracciato il percorso delle riforme, da noi fortemente volute in questa legislatura e condivise. Lo abbiamo fatto con convinzione; sono intervenuto io personalmente a nome del mio Gruppo per ribadire il nostro impegno, che si è poi trasformato in fattiva attività dei componenti della Commissione affari costituzionali e dello stesso ministro Quagliariello, esponente del mio partito, che ha dato luogo alla realizzazione di un progetto ampiamente condiviso, nel solco della mozione già approvata, in un clima di responsabilità e di collaborazione. Certamente, da parte di qualche Gruppo si possono anche non condividere alcuni aspetti, ma questo fa parte della normale logica della democrazia, guai se non fosse così. Il nostro intento rimane immutato. Vorrei rassicurare i colleghi che l'eventuale sospensione dei lavori parlamentari non inficerà né indebolirà la nostra consapevolezza

in una logica volta ad individuare percorsi alternativi, perché non intendiamo frapporci a questo disegno e a questa strategia da noi condivisa. Vi è un momento, signor Presidente, in cui le forze politiche parlamentari (perché noi in Parlamento rappresentiamo la nostra forza politica al più alto livello) avvertono il bisogno di riunirsi per discutere,

È indubbio che stiamo vivendo come partito un momento estremamente difficile. Chiediamo, sommessamente ma con convinzione, rispetto delle nostre esigenze. Concludo ribadendo

che abbiamo condiviso, condividiamo e condivideremo in questa legislatura, perché ci sta a cuore la riforma del Paese.

anche se all'ordine del giorno di oggi c'è il seguito della discussione dei disegni di legge costituzionale, ci sono le votazioni,

lavori. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari ha previsto, a maggioranza, che oggi pomeriggio l'Assemblea e le Commissioni non tengano seduta. L'esame dei disegni di legge di riforma costituzionale riprenderà domani mattina per concludersi entro domani sera, senza orario di chiusura. Conseguentemente, il previsto *question time* non avrà luogo. La Conferenza dei Capigruppo ha inoltre approvato il nuovo calendario dei lavori, che prevede sedute fino all'8 agosto, dal lunedì pomeriggio al venerdì mattina. Nel pomeriggio di lunedì 15 luglio verranno esaminate le mozioni sulla partecipazione dell'Italia al progetto dell'aereo F35. Nella restante parte della prossima settimana saranno discussi il decreto‑legge sull'IMU e ammortizzatori sociali e il disegno di legge di istituzione della Commissione parlamentare antimafia. Il calendario dei lavori delle settimane successive darà priorità all'esame dei decreti-legge presentati in prima lettura al Senato e quindi a quelli che saranno trasmessi dalla Camera dei deputati. Pertanto, nella settimana dal 22 al 26 luglio, l'Assemblea discuterà i decreti-legge in materia di occupazione e sull'esecuzione della pena; nelle settimane successive i decreti-legge, attualmente in corso di esame presso la Camera dei deputati, in materia di tutela ambiente, salute e lavoro per imprese di interesse strategico nazionale; disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia, nonché sul pagamento dei debiti degli enti del servizio sanitario. Nella seduta pomeridiana di giovedì 25 luglio, alle ore 16, si svolgeranno interrogazioni a risposta immediata, ai sensi dell'articolo 151-*bis* del Regolamento, alla presenza del Presidente del Consiglio dei ministri. Il calendario sarà integrato con le votazioni per l'elezione dei Consigli di Presidenza della Giustizia amministrativa, della Corte dei conti e della Giustizia tributaria, nonché con l'esame di documenti definiti dalla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari.

ci ritroviamo per l'ennesima volta a discutere di un'espropriazione

Tutto questo per un disegno di legge, quello costituzionale, per il quale a nostro avviso non doveva nemmeno essere avviata tutta questa macchina, e per il quale abbiamo fatto un'accelerazione al di fuori delle norme, come diceva la collega De Petris, convocando la Commissione in contemporanea all'Aula, impedendole il voto. E tutto questo, non certamente voluto da noi, oggi ci comporta una giornata inutile. Oggi è una giornata per la quale tutti noi dovremmo andare a versare un trentesimo della nostra indennità in beneficenza, come minimo,

Gruppo PdL)* che questo Parlamento non è più quello per il quale siamo stati eletti tutti quanti.

Senatore Crimi, abbiamo percepito il segno della protesta. *(Commenti)*. Oggi è una giornata particolare, allora invito al senso di responsabilità di tutti per cercare di riportare il senso di responsabilità e di equilibrio nell'ambito della nostra Aula.

Presidente, se quelli che invitano spesso gli altri a rispettare la democrazia e quest'Aula lo facessero in prima persona e con meno gazzarra forse sarebbe meglio. Vede, signor Presidente, per certi aspetti ha ragione il senatore Crimi: quest'Aula

la politica italiana sono influenzati dai grandi assenti, ma sono anche troppo spesso influenzati da grandi esterni, che volutamente sono grandi assenti che però tirano le fila della politica, anche dentro quest'Aula. *(Commenti)*. Sarebbe quindi bene che tutti avessero davvero quel senso di sobrietà che è richiesto in momenti particolarmente difficili come questo. Proprio questo senso e questa consapevolezza sottesi alla richiesta illustrata non solo con pacatezza ma anche con intelligenza e grande rispetto delle istituzioni dal presidente Schifani, sia in quest'Aula che durante la Conferenza dei Capigruppo (ed io lo ringrazio per questo)

vedremo quando la chiederete voi! Ieri facevate tante recriminazioni nei confronti degli assenti, e ci saranno stati 25 assenti tra di voi; quindi, chi è senza peccato scagli la prima pietra. *(Applausi)*. Oggi siamo in presenza della richiesta, certamente per un fatto anomalo ed esterno che non può diventare prassi e norma di questo Parlamento, di convocazione di una riunione di un Gruppo in via urgente. In funzione di questo,

ha esposto, signor Presidente, da qui all'8 agosto prefigura un'accelerazione dei tempi per poter recuperare anche quello che oggi pomeriggio non faremo. Quindi credo che debba essere segnalato all'opinione pubblica che la volontà di questo Parlamento, della maggioranza delle forze politiche e anche della maggioranza della maggioranza, non è di certo quella di fermare il tempo per fattori esterni all'attività

Presidente, ho ascoltato l'intervento del senatore Crimi: non ne condivido il contenuto, ma ho invidiato il vigore con cui lui sa intervenire in Aula. alla sua indicazione ai componenti del suo Gruppo di levarsi la giacca e la cravatta, la considero un'azione

di disprezzo volgare del Parlamento. Considero l'uscita dall'Aula dei senatori che si erano levati la giacca e la cravatta come un atto di vergogna per il loro gesto. *(Applausi Questo è il Parlamento italiano: è il Senato della Repubblica, dove i Regolamenti devono essere osservati, anche da chi non ne condivide il contenuto. Uno Stato e una Repubblica non possono vivere senza regole e chi viola queste regole assume una responsabilità grave nei confronti della democrazia. Gesti come questi, compiuti con il solo obiettivo di avere un risultato eclatante e per avere qualche fotografia sui giornali, francamente sono da disprezzare.

non debbano avvenire mai e penso che nessun Gruppo possa assumersi la responsabilità di chiedere l'interruzione del lavoro del Parlamento.

di sospensione per poter svolgere una propria assemblea politica. Questo è accaduto in passato: è accaduto perché anche noi l'abbiamo chiesto e l'Aula ce l'ha concesso.

fino a quando non avremo concluso l'esame del provvedimento costituzionale che stiamo esaminando. Considero questa sua richiesta, a cui noi abbiamo aderito (e che, quindi, ha anche condizionato il nostro voto), il riconoscimento che i lavori del Parlamento debbano continuare, che il provvedimento debba essere esaminato e concluso nella giornata di domani e che l'assemblea che il Gruppo dei senatori del PDL farà oggi pomeriggio esaurirà nel pomeriggio i suoi lavori per consentire al Senato

di essere ricevuto dal presidente della Repubblica Napolitano, perché in questo caso sarebbe chiara ed evidente una crisi di Governo.

Intanto non sto facendo una dichiarazione di voto, ma rispondo a titolo personale, e quindi ho diritto di intervenire. Vi chiedo quindi di ascoltare, perché il Presidente mi ha dato la parola. un attimo di silenzio.

tutto quello che è accaduto in quest'Aula oggi, da tutto. Ci dissociamo radicalmente dall'atteggiamento del Popolo della Libertà. Non raccontiamo chiacchiere: se si deve fare una riunione di Gruppo, non si hanno i titoli in prima pagina su tutti i giornali nazionali.

Io voglio parlare di questo, non voglio parlare di giacche e cravatte, che mi sembra - scusate se lo dico così - una vera sciocchezza. Vorrei ricordare anche ai colleghi, a quelli del Movimento 5 Stelle che se ne sono andati dall'Aula e a tutti coloro che blaterano di Aventino, che siccome le Aule parlamentari, nella storia di questo Paese, quando fu fatto l'Aventino, sono state abbandonate per una cosa gravissima, cioè l'assassinio di Giacomo Matteotti, per favore, prima di dire sciocchezze, contate fino a tre. Noi ci dissociamo da tutto.

che fa il seguito - come ha testé ricordato il presidente Zanda - ad analoghe richieste del passato e a quelle del futuro che si ripeteranno in una logica di rispetto reciproco tra forze politiche che possono nutrire diverse sensibilità. Se vi è un patrimonio da salvaguardare in quest'Aula, che è la faccia del Paese, credo esso sia quell'insieme di regole, di principi e di trasparenza fondamentali per il funzionamento della nostra democrazia.

che ha raccolto parecchi, parecchi milioni di voti in occasione delle ultime elezioni. Anche noi come voi ci sentiamo cittadini, perché lo siamo e rappresentiamo i cittadini. Siamo fieri di rappresentare quei quasi 10 milioni di elettori che ci hanno voluto in questo Senato ed hanno voluto candidato *premier* e *premier* Silvio Berlusconi. Lo sentiamo. Sentiamo di farlo. Sentiamo di riunirci e di discutere su quanto sta succedendo in questo momento nel Paese. É un dibattito che non vogliamo portare in quest'Aula, signor Presidente, perché siamo ligi al rispetto delle regole della democrazia parlamentare. Desideriamo quindi portarlo all'interno del nostro Gruppo

Mi spiace che il collega di SEL non abbia condiviso la nostra richiesta. Collega, non abbiamo bisogno di andare sui giornali per manifestare o denunziare quello che succede. Tutti succede. Tutti i giornali di oggi già ne parlano. Non vi è bisogno del nostro Gruppo perché l'opinione pubblica italiana sappia, attraverso la stampa e i programmi televisivi, che

Mi spiace poi che i colleghi del Movimento 5 Stelle abbiano abbandonato l'Aula togliendosi la giacca. Io sono in Senato, signor Presidente, dal 1996: ho fatto il senatore, il Capogruppo e ho svolto l'alto ruolo che lei sta egregiamente svolgendo in questa legislatura e devo dire che non ho mai assistito - scusate la battuta - ad un semispogliarello di miei colleghi in segno di protesta. Anche perché se siamo tenuti a un determinato decoro e ad un determinato rispetto delle istituzioni, lo facciamo proprio a tutela della dignità e della rappresentatività dei nostri stessi elettori che ci hanno portato in Parlamento, perché le istituzioni sono patrimonio di tutti. Voi siete venuti in questo Parlamento per portare le vostre idee siete venuti in quest'Aula per rappresentarle, ma non per offendere quest'Aula, perché quest'Aula è la casa di tutti gli italiani. Detto questo, signor Presidente, concludo nel dichiarare che il mio Gruppo condivide la proposta di calendario da lei esposta all'Aula